Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 29 dicembre 2016 Onorevole Presidente, informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato

Signor Presidente, onorevoli senatori, mi si chiede di informare il Senato in merito alle dichiarazioni da me rilasciate il 19 dicembre 2016 e riportate dagli organi di informazione, riguardanti il tema dei giovani che lasciano l'Italia per cercare opportunità per il loro futuro all'estero. In quella giornata ho partecipato a una serie di eventi nelle Marche. Sono intervenuto al *job day* a Pesaro, un'iniziativa promossa dal Ministero del lavoro e del nuovo disegno di politiche attive e specificamente dedicata alla promozione di opportunità di incontro diretto tra imprese, servizi, agenzie per l'impiego e giovani in cerca di occupazione. Ho poi incontrato studenti, docenti e rappresentanti dei centri e dei servizi per l'impiego

la continuità e il rafforzamento delle attività di questi enti. Inoltre, ho visitato alcune aziende della zona. Nel corso della giornata ho avuto occasione di incontrare ripetutamente i rappresentanti della stampa e degli altri mezzi di informazione che, oltre a un giudizio su questi eventi, mi hanno anche chiesto una valutazione sul fenomeno della fuga dei cervelli, ovvero dei giovani che lasciano l'Italia per cercare di realizzare i loro obiettivi in altri Paesi. Anche in ragione degli incontri svolti in quelle ore, nel corso dei quali ho dialogato con tanti giovani che si stanno impegnando per realizzare le loro aspettative nel nostro Paese, riportandone impressioni molto positive, ho risposto in modo sbagliato a questa domanda, contrapponendo lo sforzo e l'impegno di questi ragazzi che restano in Italia a quelli dei loro coetanei che scelgono un altro Paese per costruire il loro futuro. Ho sostenuto che non è giusto affermare che quelli che lasciano il nostro Paese sono i migliori e che, di conseguenza, quelli che restano hanno meno competenze e qualità degli altri. Ho aggiunto a questa opinione, che considero legittima e non offensiva, un inciso sbagliato e tale da ingenerare la convinzione di una mia insensibilità nei confronti di quei ragazzi che cercano una prospettiva lontano dall'Italia. Constatato il mio errore, ho considerato mio dovere scusarmi subito per quella espressione, anche perché molto lontana dal mio pensiero, dalla mia storia personale e dal mio modo di agire. Scuse che confermo in questa Aula parlamentare. Tuttavia, anche a conclusione della frase incriminata avevo già espresso più chiaramente il mio reale pensiero, come del resto riportato anche nel secondo dei due lanci ANSA che riferivano, quel giorno, le mie dichiarazioni. In esso, infatti, si legge testualmente: «detto questo, è bene che i nostri giovani abbiano l'opportunità di andare in giro per l'Europa e per il mondo. È un'opportunità di fare la loro esperienza, ma debbono anche avere la possibilità di tornare nel nostro Paese. Dobbiamo offrire loro l'opportunità di esprimere qui capacità, competenze e saper fare». Anche perché sappiamo che le decisioni di questi ragazzi non sono sempre una scelta obbligata, ma rispondono anche alla voglia di fare nuove esperienze e mettersi alla prova in contesti diversi. I giovani che vanno all'estero sono una risorsa importante. A tutti dobbiamo dare l'opportunità di realizzare il loro futuro nel nostro Paese o dove li portano i loro percorsi professionali e personali. Sappiamo tutti che le prospettive di lavoro dei giovani nel nostro Paese sono state fortemente compromesse dalla grande crisi iniziata nel 2008. Infatti, all'inizio di quell'anno i giovani disoccupati erano 400.000 e a marzo 2014 si era raggiunto il picco di 707.000. A novembre 2016 i giovani disoccupati sono 627.000. Un altro pesante effetto negativo è stato prodotto dalla riforma delle pensioni approvata a fine 2011 che ha fortemente innalzato l'età di pensionamento. Così come non ha aiutato la lontananza del nostro sistema di istruzione dal mondo del lavoro e dell'impresa. Su questa questione il Governo è intervenuto con l'attuazione, insieme alle Regioni, del programma europeo Garanzia Giovani che ha contribuito a ridurre di oltre 250.000 unità il numero dei giovani che non studiano e non lavorano, con l'introduzione generalizzata dell'alternanza scuola-lavoro con il potenziamento e la semplificazione dell'apprendistato e, da ultimo, con gli interventi sulle pensioni che ampliano la flessibilità in uscita e, di conseguenza, aumentano le opportunità di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In particolare, per quanto riguarda il mercato del lavoro, la disoccupazione giovanile resta a livelli preoccupanti, anche se dal marzo 2014 a novembre 2016 è diminuita di 3,5 punti. C'è poi, naturalmente, anche un tema di qualità del lavoro. Il nostro impegno è stato ed è quello di aumentarne la stabilità e ridurne la precarietà. Con la riforma del mercato del lavoro abbiamo abolito una serie di contratti con forti connotati di precarietà, come i contratti di collaborazione a progetto e le associazioni in partecipazione. Abbiamo più rigorosamente definito il confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo per combattere il fenomeno delle false partite IVA. I dati ISTAT confermano che l'incremento degli occupati è largamente ascrivibile al lavoro dipendente stabile. Infatti, dei 593.000 occupati in più rispetto a marzo 2014, 442.000 sono lavoratori permanenti. Su questo tema oggi è aperta una riflessione sull'utilizzo dei *voucher*. Colgo l'occasione di questa comunicazione per ribadire, come già peraltro affermato dal presidente del Consiglio Gentiloni e in relazione alle prime evidenze tratte dall'analisi dei dati di monitoraggio sull'uso dei *voucher*, che il Governo considera necessaria una revisione di questo strumento, al fine di riportarlo alla funzione per la quale era stato disegnato, ovvero di dare copertura previdenziale e assicurativa alle attività occasionali, portandole fuori dal lavoro nero. Mi sia consentita, ancora, una considerazione finale. Intorno alle dichiarazioni da me rilasciate il 19 dicembre, insieme alla comprensibile e giustificata polemica politica, si è sviluppata, in particolare sui *social media*, una campagna di insulti e minacce che non ha colpito solo me, ma ha coinvolto la mia famiglia: mia moglie e mio figlio. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino e hanno espresso a me e alla mia famiglia la loro solidarietà per questi episodi che, al di là della preoccupazione e del disagio che provocano alle persone direttamente coinvolte, non possono trovare alcuna giustificazione e allarmano perché testimoniano un clima di tensione. Sono episodi che non hanno nulla a che vedere con le critiche e le contestazioni, anche aspre, che si mantengano nell'ambito di un confronto civile e rispettoso. In conclusione, mi auguro di avere corrisposto puntualmente alla richiesta di informativa che mi era stata proposta e di avere chiarito il mio pensiero sull'argomento in discussione. *(Applausi

colleghi, credo che dal momento che siamo chiamati a discutere di un problema estremamente serio, quello dell'occupazione in Italia e, in particolare, della disoccupazione giovanile, dovremmo essere tutti più consapevoli che questi temi meritano la massima serietà e respingere la tentazione di affrontare la discussione sull'onda di strumentalizzazioni politiche, magari di precedenti voti referendari o di dichiarazioni che ha fatto il Ministro. Trovo invece utile e necessario che si analizzi il lavoro svolto finora dal Ministro e si valuti se è la persona giusta per occuparsi di problemi così grandi e urgenti, partendo da una domanda fondamentale: quale modello di mercato del lavoro vogliamo avere in Italia? O, meglio ancora, quale modello è più attrattivo per i giovani?

Verso Paesi dove il posto di lavoro è maggiormente tutelato che in Italia? Verso economie stagnanti, poco produttive, chiuse, nelle quali il merito e la competizione sono considerati principi nemici dei diritti dei lavoratori? Ci dichiariamo indignati per i tanti giovani che lasciano l'Italia, ma neppure ci preoccupiamo allora di guardare cosa vanno cercando. Stati Uniti, Inghilterra, la stessa Germania e tutte le nuove mete a disposizione di chi varca i confini nazionali, non attirano certo i nostri giovani grazie ad una maggiore rigidità del mercato del lavoro.

Come i dati e le ricerche testimoniano, la correlazione tra flessibilità e maggiore occupazione è pressoché nulla. Dico però che i nostri giovani scelgono di lavorare in Paesi in cui non si contesta la flessibilità del mercato del lavoro perché essa è il frutto di una cultura

Ciò che può fare la differenza in Italia non sono norme migliori che regolino il mercato del lavoro, ma un approccio pragmatico e *post* ideologico che porti a scegliere convintamente e coerentemente il modello che coniuga flessibilità e sicurezza per il lavoratore (perché di flessibilità mi pare che ve ne sia anche troppa, oltre alla mancanza di occupazione) con la sicurezza di trovare un impiego che veramente interessi la persona. creare una normativa più certa e sicura che attiri investimenti nel nostro Paese, perché questo continuo cambiare delle regole certamente non ci rende credibili. È di ieri, nuovamente, il dato secondo cui la disoccupazione giovanile ritornata al 40 per cento. Come più volte si dice, andare all'estero deve essere una scelta, un'opportunità, dettata dalla voglia di andare a fare nuove scoperte, non deve essere una necessità perché qui non si riesce a far valere il proprio merito e il proprio sapere.

Signor Ministro, per il ministro Padoa Schioppa i giovani erano bamboccioni, per la ministra Fornero erano troppo esigenti e pretenziosi, mentre lei, signor Ministro, parlando dei giovani che lasciano l'Italia per trovare lavoro all'estero, arriva a dichiarare che conosce «gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo Paese non soffrirà a non averli più fra i piedi». In un qualsiasi altro Paese, dopo simili esternazioni chiunque avrebbe l'obbligo di dimettersi. Ma a bocciare le vostre politiche e quelle del suo Governo, signor Ministro, ci pensano gli elettori, i quali, in ogni occasione in cui vengono chiamati alle urne, dimostrano come questa maggioranza non rispecchi affatto la società e sia scollata dalle problematiche reali.

Mettendo da parte le sue infelici dichiarazioni, dovremmo concentrarci sul perché ci siano questi dati, sul perché le vostre politiche occupazionali e sul lavoro non abbiano funzionato e sul perché i nostri ragazzi debbano sperare in un futuro migliore solo lasciando la nostra terra. Vorrei dirle, signor Ministro, che decidere per i nostri giovani di lasciare le proprie famiglie e i propri affetti, non sempre risulta una scelta libera e spensierata. No, troppo spesso risulta essere una fuga obbligata, un'ultima possibilità. La disperazione di questa scelta non è solo quella dei ragazzi che salgono sul primo volo diretto magari in un qualsiasi Paese europeo, ma è la disperazione e la preoccupazione di migliaia di genitori che arrivano al punto di sentirsi colpevoli per non aver saputo dare al proprio figlio o alla propria figlia una prospettiva di vita nella loro Patria. Il compito del Governo, quello che lei rappresenta, dovrebbe essere quello di trovare soluzioni adeguate per dare e ridare speranza alle nuove generazioni, invece di rilasciare dichiarazioni che un Ministro, secondo me, non può permettersi di fare. Se lei, signor Ministro, vuole veramente che le sue scuse vengano accettate, metta in atto politiche sociali idonee. Inizi a riconoscere i fallimenti causati dal famigerato *jobs che non ha prodotto i risultati annunciati nonostante le ingenti risorse messe a disposizione e che non ha saputo incidere fattivamente sul mercato del lavoro, aumentando la precarietà per i lavoratori e non offrendo alle aziende strumenti adeguati per investire ed assumere. Si confronti, signor Ministro, anche con le opposizioni. Iniziamo a cambiarlo, questo futuro, lo dobbiamo ai nostri giovani. Si adoperi, signor Ministro, affinché i cervelli, invece di fuggire, restino nel nostro Paese, dove hanno studiato, si sono formati e dove - ne siamo tutti certi - vorrebbero sicuramente restare. Caro Ministro, lei non deve dimettersi, anche perché non lo fecero né Padoa Schioppa, né la Fornero, dopo aver rilasciato affermazioni poco opportune sui nostri ragazzi. Ma dia risposte ai nostri ragazzi, ai tanti che nemmeno cercano più un'occupazione, perché stanchi, demotivati e rassegnati. Le assicuro, signor Ministro, che guardare negli occhi un ragazzo che non sogna più, a cui abbiamo tagliato tutte le aspettative, è come vederlo morire lentamente. E questo è inaccettabile. Il diritto al lavoro è un principio sancito nella nostra Costituzione, quella che i cittadini, nell'ultimo voto referendario, hanno difeso e protetto e noi dobbiamo ripartire da quel diritto, dagli articoli 1 e 4 della nostra Carta costituzionale, che forse in pochi hanno letto adeguatamente. Signor Ministro, ridiamo speranza e futuro a questo Paese e ai nostri giovani.

Ministro, parliamo solo di quanto tocca lei e delle sue responsabilità: i dati di oggi, che non risalgono a un anno fa ma che abbiamo letto questa mattina, dicono esattamente il contrario, c'è una disoccupazione arrivata al 12 per cento e non può essere letta con il dato che ci ha dato lei, di qualche mese fa, che sembrava tendenzialmente di segno contrario.

la verifica, dopo tre anni. Era inutile dire che vi sono state assunzioni, perché ora si manifesta tutto l'aspetto negativo: sono finiti gli incentivi, le imprese non hanno più interesse e non si assume più nessuno e i dati purtroppo, non ne siamo felici, ma dobbiamo leggerli per quelli che sono. Ministro, noi sappiamo delle cose e ci chiediamo: ma il Governo lo sa? Prendiamo quelle politiche sciocche, fatte per i giovani, come i 500 euro dati ai maggiorenni: sapete che fine hanno fatto?

Credo abbia letto anche lei il dato dei patronati svizzeri: il suo Ministero eroga tra i 35 e i 40 milioni l'anno. Siamo sorpresi che un direttore del patronato CGIL-INCA di Zurigo si sia potuto appropriare di cifre che sorpassano i dieci milioni e infatti il tribunale di Zurigo, nel 2015, lo ha condannato a nove anni di carcere.

che evidenziava queste storture: non si è fatto assolutamente nulla. Signor Ministro, lei ha annunciato che vi saranno delle ispezioni,

dove mettere i ricoverati Ma la sanità non si gestisce in modo ragionieristico, la sanità va gestita

Mi fermo qui. che decidono di arrangiarsi senza chiedere niente allo Stato, come hanno fatto i migranti nell'Ottocento e all'inizio del Novecento che hanno deciso di trovare la loro strada, devono sentirsi anche umiliati da un rappresentante del Governo? Questa è la del Governo? Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Ci siamo sentiti in dovere di firmare - non è un'iniziativa nostra, ma dei colleghi di SEL - una chiamata di responsabilità diretta da parte sua. Non sarebbe male se ogni tanto, all'interno del Governo, quando succedono queste cose, qualcuno dicesse: «non mi giustifico, ho delle colpe, ho fatto degli errori», come si fa in tutti i Paesi normali e democratici. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà. signor Ministro, ieri sono stato invitato a una trasmissione televisiva e non ho potuto fare a meno di pensare a lei, La trasmissione si è aperta infatti con i dati ISTAT sull'occupazione. Poi c'è stato un servizio sui Comuni in *default*

e giovani che sono senza lavoro. Infine, è stato trasmesso un servizio sull'ospedale di Nola. Oggettivamente, il nostro Paese si trova in una situazione di forte difficoltà. A prescindere da tali immagini, credo che su questo possiamo convenire. Io le confesso, signor Ministro, che il suo linguaggio mi è simpatico, anche perché sono un oppositore del politicamente corretto. Però le devo altresì dire che c'è un senso delle istituzioni che dovrebbe portare a una considerazione del tempo storico che stiamo vivendo. Quando non si occupa un ruolo istituzionale, ci si può esprimere come si vuole. Nel momento in cui si accetta quella che è sì una carica, ma a volte è anche un peso, bisogna adeguarsi a quello che il ruolo istituzionale richiede. Lei, signor Ministro, questo non l'ha fatto. Lei ha offeso i nostri giovani costretti ad andare all'estero, ma ha anche mostrato di non aver compreso, a mio avviso, il fenomeno dell'occupazione in una società globalizzata. Lei ha proposto un'immagine autarchica

quello che noi dovremmo garantire al nostro Paese in questo momento storico è che alcune intelligenze possano andare all'estero, ma altre possano venire qui; e che l'Italia, per la quale l'intelligenza è sempre stata un fattore di sviluppo, non abbia una perdita secca per una situazione nella quale l'esportazione diventa una necessità e la circolarità del lavoro si blocca anche perché evidentemente chi dovrebbe comprendere questo fenomeno non lo comprende. Questa sarebbe una perdita secca per il nostro Paese. ha esordito in maniera dignitosa dicendo «ho sbagliato» e chiedendo scusa. A volte, tutto ciò può essere anche accompagnato da

un'offesa, non è un mostrarsi debole, ma molto spesso è un mostrarsi forte e considerare il proprio incarico come un impegno nei confronti del Paese da portare avanti finché non si sbaglia troppo. È una prova di sensibilità che noi ci augureremmo perché sarebbe anche un cambiamento di clima e di segno rispetto a quello che abbiamo visto nel nostro più recente passato.

per ignoranza, ma ha sbagliato e quel chirurgo non può più fare il primario di quell'unità operativa, perché non ha più nulla da insegnare.

aveva fatto un grande lavoro, eppure ha dovuto lasciare. Emblematica è la mozione di sfiducia da parte dell'attuale ministro Franceschini nei confronti di Sandro Bondi per un piccolo crollo a Pompei; dopodiché negli ultimi tre mesi è crollato praticamente tutto: addirittura c'è un'indagine della procura sui crolli al tempio di Venere, alla necropoli

a quel chirurgo che non ha mai sbagliato; ma nel momento stesso in cui asporta il rene sbagliato al posto di quello sano non può più dirigere quell'unità operativa. Le chiediamo quindi di toglierci dall'imbarazzo e di fare la scelta che noi riteniamo più giusta, che non è quell'applauso che è venuto da alcuni banchi, perché quello ovviamente non lo merita, in quanto quelle frasi sono da respingere e da condannare. Accettiamo le sue scuse e la sua ammissione di responsabilità,

Signor Presidente, signori senatori, oggi non avrei parlato, ma ho ascoltato l'intervento del signor Ministro, come del resto negli anni scorsi ho ascoltato anche quanto ci ha detto ripetutamente in materia di lavoro: se i dati erano positivi era merito del Governo, altrimenti non se ne parlava.

In realtà, in uno scenario economico e sociale che non è più solo internazionale ma anche globale, la complessità dei fenomeni è enorme e la possibilità di stabilire collegamenti così puntiformi tra alcuni dati generali e l'azione particolare di un Governo è semplicemente assurda. Inoltre, lo stesso vale per l'azione del Governo: pensare che il Governo determini tutti questi fatti, come il PIL o il lavoro, è francamente fuori da ogni logica. Per questo effetto di complessiva confusione nell'ordine dei fattori io credo che lei non debba essere privato della fiducia per aver commesso o detto alcune cose, ma per non averle comprese.

per fin troppo tempo hanno occupato il dibattito pubblico e a nome del mio Gruppo non posso che esprimere apprezzamento per quello che il Ministro ha detto. Come Gruppo per le Autonomie abbiamo giudicato tali affermazioni inopportune quando sono state rese pubbliche; confermiamo tale giudizio, mentre riconosciamo al ministro Poletti l'onestà intellettuale e politica di aver riconosciuto la necessità di correggere profondamente quanto affermato. Del resto le dichiarazioni del Ministro, che senz'altro potremmo definire quantomeno avventate, potevano ben più facilmente essere contraddette dalle molte iniziative che questo Governo, come anche di quello che lo ha preceduto della maggioranza che ha sostenuto entrambi, hanno messo in atto per imprimere dei cambiamenti importanti nel mercato del lavoro italiano proprio nei confronti di quei giovani che soffrono di più le rigidità del sistema. In un tempo in cui i dati statistici (basti vedere le ultime rilevazioni che l'ISTAT ha rilasciato proprio ieri) ci restituiscono l'immagine di un mondo del lavoro che ha sostanzialmente tenuto alla crisi economica, ma che ancora stenta a riprendere quota, occorrerebbe il coraggio di riconoscere queste novità, di non rimettere in discussione i fondamenti e anzi, laddove sarà possibile, di fare ulteriori passi avanti nella direzione intrapresa. Per questo, a nome del Gruppo Per le Autonomie, desidero rivendicare alcune di queste importanti iniziative proprio alla presenza del Ministro stesso, facendo solo due riferimenti, che sono anche di grande attualità, dato che se domani la Corte costituzionale dovesse dichiararne 1'ammissibilità, potrebbero essere sottoposte al giudizio popolare tramite *referendum*. Il primo riferimento riguarda in generale il *jobs act* (e la parziale abolizione dell'articolo 18); il secondo la regolazione dell'uso dei *voucher*. Nel primo caso si è voluto semplificare l'impianto regolatorio del mercato, sottraendolo ad alcune rigidità e a un eccesso di burocratizzazione che troppo spesso ha penalizzato lavoratori e imprese inibendo la propensione ad assumere. In un contesto come quello italiano, fortemente sindacalizzato e soggetto ad una conservazione corporativa che difficilmente si può rintracciare in altri Paesi occidentali, il *jobs act* ha rappresentato una riforma che persino Francia o Germania hanno apprezzato e in parte anche ripreso. Il secondo tema, signor Ministro, sono i *voucher*: un argomento che sta molto a cuore a tutto il mondo del lavoro del mio territorio, la provincia di Bolzano - come è stato accennato poc'anzi e di cui rivendichiamo senza inibizioni l'efficacia tanto da chiedere a lei, signor Ministro, di non apporre alcuna modifiche ad una legislazione che già ha subito un irrigidimento che non era auspicabile. Come mostrano i dati recentemente resi dagli enti competenti, che si riferiscono in particolar modo al nostro territorio, l'utilizzo dei *voucher,* soprattutto in agricoltura e nel turismo, ha dato la possibilità di attivare nuove posizioni lavorative facendo occupazione in modo legale.

porto sempre l'esempio della realtà in cui opero e che rappresento - non solo l'attivazione dei contratti a tempo determinato è aumentata ma ad aumentare è stata soprattutto la cosiddetta occupazione occasionale che in passato non si faceva: non si riusciva a farla perché non esistevano strumenti per legalizzare forme di lavoro che non potevano essere inquadrate né nel tempo determinato né in quello indeterminato. Per queste ragioni, signor Ministro, le esprimo la nostra solidarietà.

*(Misto-SI-SEL)*. Signor Ministro, noi di Sinistra Italiana, insieme ad altre forze politiche, abbiamo presentato una mozione di sfiducia

Ha parlato di qualità del lavoro; evidentemente o lei non vive in Italia oppure mente spudoratamente, perché, al di là del fatto che il lavoro non c'è, quel poco che c'è della qualità non sa proprio cosa farsene, la qualità del lavoro non esiste più. Forse a lei sfugge il fatto che ormai il lavoro in Italia è ridotto a *voucher* (121 milioni

scusare con i nostri giovani. Penso che in un Paese democratico le scuse vadano accettate se sono sincere, signor Ministro. Forse a lei sfugge

alle persone che ne hanno bisogno e sarebbero rimasti in Italia, sarebbero stati rimessi in circolo nell'economia. Lei ha regalato 20 miliardi di soldi pubblici

aleggiano le mozioni di sfiducia presentate da alcuni Gruppi della minoranza. Sono stato avversario e concorrente di Giuliano Poletti,

Poletti, come ovvio, non nasce Ministro; ha una sua storia che parla per lui e che non è né oscura né contraddittoria.

Sono testimone diretto delle tante dichiarazioni di Poletti e della passione con la quale ha sostenuto e portato ad esempio cooperative giovanili e l'impegno delle nuove generazioni nelle imprese. Le mie idee non collimavano ieri e non collimano oggi del tutto con le sue, ma ho sempre apprezzato l'onestà intellettuale e personale, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

non ha offeso i giovani, come ha detto il senatore Quagliariello; nel modo più assoluto. Lei non ha detto che i giovani che lasciano il nostro Paese sono un peso di cui liberarsi. Chi ha fortemente strumentalizzato e criticato le sue parole si è soffermato solo sulle prime righe della sua dichiarazione.

«Dobbiamo offrire l'opportunità ai giovani di esprimere qui (ossia in Italia) capacità, competenza e saper fare». è questo se non il richiamo al sistema Italia per rendere più efficiente e competitiva la nostra impresa in modo da assorbire occupazione e, ovviamente, sempre più quella giovanile? Lo spirito delle dichiarazioni che oggi lei ha reso dimostrano il suo pensiero e i suoi intendimenti, al di là delle strumentalizzazioni che ho ancora sentito in quest'Aula. Vogliamo parlare dei giovani? Vogliamo parlare dei giovani che vanno all'estero? Vogliamo parlare della cosiddetta fuga dei cervelli? Ci soffermeremo

non consente lo svolgimento del *referendum* questo non è corretto, né giusto. Il Paese ha bisogno di confrontarsi nuovamente

che l'informativa resa in Aula dal ministro Poletti abbia messo fine alle polemiche strumentali. Signor Ministro, le esprimiamo anche la nostra solidarietà personale e di Gruppo

Signor Ministro, lei oggi si presenta qui con il capo cosparso di cenere e chiede scusa per una sua esternazione infelice. Ne prendiamo atto. Lei fa

lei parte con la crisi del 2008, la riforma delle pensioni del 2011 e lo scollamento tra scuola e impresa, perché c'è l'urgenza di creare dei giovani che abbiano delle capacità, delle competenze e del saper fare. Per noi, invece, bisogna creare degli adulti che sappiano essere cittadini attivi e partecipi in questa società, i quali sappiano quindi Poi continua raccontandoci - e qui sta lo scivolone la sua favola, la favola di un Ministro nel Paese delle meraviglie. Io, invece, la vorrei risvegliare da questa favola perché in questo mondo delle meraviglie che lei ci ha raccontato snocciolando qualche dato, in realtà, non vivono tanti

attestandosi al 39,4 per cento, e il tasso di disoccupazione generale è all'11,9 se non consideriamo gli inattivi perché, Ministro, tante persone hanno perso lo spirito e la voglia di cercare lavoro, sono frustrate e depresse perché non vedono prospettive. Allora, se noi aggiungiamo queste persone e le contiamo arriviamo ad un tasso di disoccupazione che sfiora il 20 per cento. Il mondo del lavoro non è certo migliorato, mi scusi, con le sue politiche perché il *jobs act* ha fatto tutto tranne

Gli sgravi contributivi che erano stati previsti per favorire le assunzioni a tempo indeterminato, mi scusi Ministro, sono serviti a creare una narrativa, una bolla una bolla occupazionale che fa parte solo della vostra narrativa politica più che di dati reali, una narrativa politica, uno *slogan* che voi avete utilizzato variamente per tentare di portare a casa altri altri obiettivi politici che non fossero quello di dare veramente stabilità e di combattere la precarietà in questo Paese.

autoreferenziale che in questa legislatura ha dimostrato di avere maggiore attenzione per gli interessi delle *lobby*, delle banche, delle assicurazioni e dei propri interessi in campo piuttosto che per varare veramente delle politiche a favore dei giovani e meno giovani per non subire la precarietà quotidiana la precarietà quotidiana non solo materiale ma anche emotiva, che deriva dal non poter contare su un lavoro o sul potersi ricollocare in un mondo del lavoro veramente flessibile e che funzioni. Abbiamo il 28,7 per cento degli italiani a rischio povertà o esclusione sociale. Il reddito di cittadinanza, la nostra proposta, giace da due anni e più nella Commissione di competenza perché voi non volete ragionare e siete ciechi su questo. per cento delle persone dichiara di non potersi permettere una settimana di vacanza, il 17 per cento di non poter riscaldare adeguatamente le proprie case, l'11,8 cento delle persone dichiara di non riuscire a fare un pranzo adeguato e il 15 per cento delle persone dichiara di avere avuto arretrati per mutui, affitti o bollette. Chiudono 390 imprese al giorno e 11 milioni di persone rinunciano alle cure e questo perché voi avete portato avanti delle politiche, e lei ha portato avanti delle politiche nel mondo del lavoro che non solo hanno tradito le attese dei giovani e dei loro genitori, ma hanno tradito anche i principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale perché l'articolo 3 impone alla Repubblica di portare avanti delle politiche che assicurino

a chi governa di garantire il diritto al lavoro, perché è anche (e non solo) attraverso il lavoro che si attua lo sviluppo della persona umana. Allora, caro Ministro, spero di rivederla in quest'Aula a presentare misure concrete per fare in modo che i giovani non si sentano abbandonati, ma si sentano accompagnati e ascoltati da un Governo che è in perfetta

che il vero senso della politica sia l'umanità, non toccherò temi politici e mi soffermerò solo sul senso reale e sostanziale delle sue dichiarazioni. Signor Ministro, lei ha affermato che l'Italia non soffrirà a non avere più tra i piedi le persone che se ne sono andate all'estero: è testuale. Allora, signor Ministro, le vorrei dire una cosa: lei sa che questo Paese è stato percorso per anni dall'emigrazione e lei sa quanta attenzione la nostra Costituzione e noi stessi prestiamo agli italiani all'estero, tanto da consentire loro il diritto di voto. Davvero lei pensa, signor Ministro, che la nostra Italia non soffrirà o non ha sofferto a non avere più tra i piedi Renato Dulbecco, Rita Levi Montalcini o il nostro collega, senatore Carlo Rubbia, che furono costretti ad andare a lavorare all'estero e lì, attraverso i loro studi e le loro ricerche, raccogliere il frutto di un premio Nobel?

Vede, signor Ministro, sia lei che il senatore Marino, nel ripetere le frasi che lei ebbe a pronunciare, vi siete soffermati su un punto del secondo periodo e avete entrambi saltato un sue dichiarazioni che rappresenta esattamente il suo pensiero e la sua inadeguatezza a fare il Ministro: dobbiamo dare loro l'opportunità di tornare a casa. No, signor Ministro; un Ministro del lavoro deve lavorare per dare ai giovani italiani l'opportunità di poter lavorare qui in Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Signor Ministro, diciamoci le cose come stanno: i nostri figli, salvo quelli che, per le loro particolari specializzazioni, hanno necessità di andare a lavorare all'estero, all'estero non ci vanno. Non ci vanno perché qui hanno protezione familiare e hanno le famiglie che li supportano. In altri termini, quei giovani che vanno fuori sono giovani senza protezione familiare che vivono il dramma di una selezione non meritocratica che è propria di questo Paese

grave dramma che c'è in questo Paese. Non è solo e tanto quello dei giovani che sono costretti ad andare a lavorare all'estero, quanto quello del distacco dalle famiglie, da tutte quelle famiglie che sanno o immaginano di sapere di avere dei giovani che non sono dei "pistola" e non sono i peggiori di tutti, ma sono dei giovani che non riescono a lavorare in questo Paese e sono costretti ad andarsene via. E lei, in ordine a tutto questo, cosa ci dice? Ci dice che l'Italia non si preoccuperà a non averli più tra i piedi. Io credo che le sue scuse non siano accettabili e mi chiedo una cosa. Lo dico con molta franchezza; l'ho detto in un comunicato stampa immediatamente dopo le sue dichiarazioni e lo ripeto qui in Aula. Lei ritiene davvero che le sue scuse possano essere accettate dai familiari di Valeria Soresin, di Fabrizia Di Lorenzo, di Giulio Regeni, tutti e tre andati a lavorare all'estero perché non avevano avuto la possibilità di trovare lavoro qui in Italia? In conclusione, signor Ministro, lei ha la sua età e la sua esperienza: prenda atto della situazione, prenda atto del fatto che le sue dichiarazioni non possono essere scusate

noi prendiamo atto delle scuse del Ministro in questa prestigiosa Aula del Senato. Un atto di scusa è un atto di umiltà e di forza nello stesso tempo, e anche di grande responsabilità. Per noi il caso è chiuso. Ma, per affrontare questi temi, noi abbiamo bisogno di operazioni di verità. Intanto, per affrontare il tema della cosiddetta fuga dei cervelli, credo che il Ministro non abbia detto una cosa sbagliata quando ha detto

In primo luogo, noi viviamo oggi in un mondo che offre molte più opportunità rispetto alle generazioni precedenti. Quindi la fuga dei cervelli dovremmo ribattezzarla come una grande opportunità. Chi sceglie di fare un'esperienza all'estero è più libero di farla rispetto al passato. In un mondo globale, sono molte di più le *équipe* internazionali, soprattutto in campo scientifico, ed è fondamentale la collaborazione fra talenti. In Italia ci sono molti esempi di eccellenza: abbiamo cartelline piene di nostri giovani che vengono premiati e di nostri centri di eccellenza che sono all'avanguardia nel mondo.

anni. Pensiamo a quanto è cambiata la storia delle generazioni. Il mondo in cui viviamo è un mondo globale, in cui i nostri figli hanno il sapere in tasca ed hanno accesso al mondo. Questo è. E quando il senatore Quagliariello parla di circolarità del lavoro, si riferisce esattamente a questo. In secondo luogo, per chi vuole tornare in Italia, ci deve essere qui una politica pubblica che aiuti il rientro dei nostri giovani che scelgono di rientrare in Italia. Nella legge di stabilità abbiamo inserito un aiuto sostanzioso, dal punto di vista fiscale, per i nostri ragazzi (i cosiddetti "cervelli in fuga") che hanno voglia di tornare in Italia. nostro impegno è come tutti possono accedere a questo mondo aperto, e quindi costruire una società in cui ci siano pari opportunità di accesso, e come il nostro Paese diventa attrattivo (sviluppare e creare posti di lavoro). Ricordo che nella legge di stabilità è contenuto un pacchetto di misure, che non vi è mai stato prima (Industria 4.0), per rendere il nostro Paese attrattivo.

Ma la politica pubblica vera è quella che rafforza e mira a sostenere le competenze dei giovani in un mondo aperto e globale. Quindi, il tema della politica oggi è costruire opportunità in Italia per chi vuole rimanere e sviluppare un sistema che riesca ad attrarre anche chi vuole entrare nel nostro Paese. osservazione sui dati, come ho fatto già in altre occasioni. Noi possiamo dividerci, maggioranza e opposizione, sulla qualità e sui tipi di interventi da fare sul lavoro,

annuale degli occupati è indice del fatto che andiamo verso una stabilizzazione dell'occupazione, anche in presenza di una notevole crisi economica, pur nella flessione dei dati occupazionali del mese di novembre. della disoccupazione giovanile indica la diminuzione degli inattivi. I nostri giovani, cioè, hanno più fiducia nel presentarsi e nel cercare lavoro.

una vera politica attiva, perché solo così noi potremo intercettare il senso di scoraggiamento e di solitudine dei nostri giovani. Questa è una politica di verità, e decidere misure pubbliche per aiutare i giovani fa parte della responsabilità di tutti. Concludo dicendo che non è tollerabile, né giustificabile, né pensabile l'attacco che il Ministro e la famiglia del Ministro hanno subito in queste ore. dal Gruppo PD)*. I cittadini e le cittadine, soprattutto i più giovani, hanno bisogno di soluzioni e non di un clima di odio e violenza. E, per cortesia, è responsabilità di tutti noi, maggioranza e opposizione, stare attenti alle parole che usiamo qui, al linguaggio, perché noi dobbiamo essere per primi di esempio per i nostri ragazzi che si affacciano al futuro.

la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Albertini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo alla relatrice, senatrice Filippin, se intende intervenire.

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, la fattispecie in questione inerisce al procedimento penale n. 7061 del 2013 per il delitto di calunnia aggravata, di cui al combinato disposto degli articoli n. 368 e 61, n. 10, del codice penale. Le indagini relative a tale procedimento a carico del senatore Albertini si sono concluse il 26 giugno 2014, come risulta dall'avviso di conclusione delle indagini, in pari data, trasmesso dalla procura di Brescia al Senato con lettera in data 13 agosto 2014. All'origine di questo procedimento vi è l'esposto inviato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia dal senatore Gabriele Albertini, all'epoca parlamentare europeo, sull'operato del dottor Alfredo Robledo. Prima di proseguire nell'esame della vicenda connessa al procedimento penale n. 7061 del 2013, su cui l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi, è necessario dare conto della storia complessa e articolata che ha visto confrontarsi ripetutamente, in varie sedi e con vari ruoli, il già sindaco di Milano ed europarlamentare, Gabriele Albertini, poi senatore, e il dottor Alfredo Robledo, allora procuratore aggiunto a Milano. La prima fase attiene al procedimento civile avanti il tribunale di Brescia (n. 17851 del conseguente alla citazione in giudizio dell'allora eurodeputato Gabriele Albertini da parte del pubblico ministero Alfredo Robledo, in relazione all'intervista rilasciata alla testata giornalistica «Il Sole 24 Ore» intitolata: «Il processo derivati e l'ira di Albertini»,

per diffamazione avanti il tribunale di Brescia (n. 17851 del 2012). In relazione a tale procedimento, il senatore Albertini, all'epoca parlamentare europeo, presentava la richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità, ma questa richiesta veniva respinta dal Parlamento europeo in data 21 maggio 2013. Uguale destino aveva la richiesta di riesame del 17 luglio 2013, respinta dal Parlamento europeo il 24 febbraio 2014. Il 7 agosto 2014 il senatore Albertini investiva quindi il Senato, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, della questione di insindacabilità delle opinioni espresse nelle interviste che avevano originato la predetta causa civile. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiamata all'esame il 3 settembre 2014, proponeva all'Assemblea del Senato di dichiarare la propria incompetenza ritenendo sussistere la competenza del Parlamento europeo. Ciò in quanto il senatore Albertini, all'epoca di tali interviste (2011), era membro dell'Europarlamento e per essere stato quest'ultimo investito del problema anche in sede di riesame. Il 4 dicembre 2014 l'Assemblea del Senato approvava la proposta della Giunta *de qua* dichiarando la sua incompetenza a deliberare perché l'interessato non rivestiva la qualifica di senatore all'epoca dei fatti. La seconda fase invece attiene ad un procedimento penale (n. 7061 del 2013) pendente presso il tribunale di Brescia per calunnia aggravata. Come si ricordava, all'origine di questo procedimento vi è un esposto inviato in data 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia dal senatore Gabriele Albertini, all'epoca parlamentare europeo, sull'operato del dottor Robledo. Anche per tale procedimento penale, il senatore Albertini, in data 28 luglio, inoltrava al Parlamento europeo la richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità. Contestualmente, però, il 29 luglio 2014, il senatore Albertini richiedeva al Presidente del Senato, sempre per il suddetto procedimento penale, di investire il Senato circa la sua insindacabilità delle opinioni espresse. Il 25 marzo giungeva la decisione del Parlamento europeo, che confermava le precedenti decisioni del 21 maggio 2013 e del 24 febbraio 2014, riferite però al procedimento civile, quindi statuiva sulla non difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini in relazione al procedimento penale. La motivazione addotta dal Parlamento europeo era non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di un nesso diretto ed evidente tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari Con nota del 13 giugno 2016, il senatore Albertini presentata quindi una nuova istanza alla Giunta del Senato, interamente sostitutiva della precedente, in cui richiedeva, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione per il procedimento penale l'insindacabilità delle opinioni espresse. In essa il senatore Albertini mutava radicalmente la richiesta affermando, diversamente da prima, la competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato anche per la sua allora qualità di parlamentare europeo, e chiedeva di far valere l'insindacabilità delle opinioni espresse in quanto compiute nello svolgimento specifico della sua attività. Come detto fino a questo momento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e quest'Assemblea si erano già espresse sulla questione relativamente al giudizio civile n. 17851 del 2012 per diffamazione, pendente sempre davanti al tribunale di Brescia. Stante la diversità dei procedimenti - civile il primo, penale il secondo - originati da fatti diversi (interviste nel primo caso ed esposto al Ministro della giustizia nel secondo), si ritiene non sia invocabile il principio del *ne bis in idem*. Così ricostruita la complessiva storia conseguente le dichiarazioni rese dal senatore Albertini, sussistono argomenti in forza dei quali si ritiene che le opinioni espresse dal senatore possano considerarsi coperte dalla guarentigia dell'insindacabilità. Innanzitutto, la questione della competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e quindi dell'Assemblea è, in sostanza, quella della sussistenza dei presupposti scriminanti le presunte condotte calunnatorie del senatore Albertini. Come ricordavo, all'origine di questo procedimento vi è l'esposto inviato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia dal senatore Albertini, all'epoca incontestabilmente parlamentare europeo, sull'operato del dottor Robledo. Tuttavia, questo esposto ha rappresentato soltanto un capitolo di una lunga sequela di atti e di reazioni, che ha visto il magistrato e il senatore confrontarsi ripetutamente, con esternazioni, denunce, querele ed esposti. Ne rammento solo i più significativi, dando conto anche della loro successione temporale: in data 22 ottobre 2012, come ricordavo, Gabriele Albertini, allora parlamentare europeo, inviava al Ministro di giustizia l'esposto più volte citato. Il 24 febbraio 2013 Gabriele Albertini veniva eletto senatore. Il 27 marzo 2013 il dottor Robledo denunciava il senatore Albertini per quanto dichiarato nell'esposto del 22 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 368 del codice penale e 61, n. 10, dello stesso codice penale ovvero per calunnia aggravata. In data 4 luglio 2013 il senatore Albertini rinnovava l'esposto al Consiglio superiore della magistratura, cui seguiva, in data 20 settembre 2013, la trasmissione del suddetto esposto - sempre lo stesso - procuratore generale presso la Cassazione. Il 29 gennaio 2014 il senatore Albertini presentava un'interrogazione al Ministro di giustizia, sempre con il medesimo contenuto. In assenza di risposta, l'interrogazione veniva riproposta in data 10 giugno 2014. In data 18 giugno 2014 il Ministro di giustizia rispondeva ad entrambe le interrogazioni. data 26 giugno 2014 si concludevano però le indagini, per cui la procura di Brescia trasmetteva l'avviso di conclusione delle stesse. La richiesta di rinvio a giudizio del senatore Albertini da parte del pubblico ministero di Brescia è del 23 ottobre 2014. Questa è però solo una parte. Il senatore Albertini risulta aver svolto interventi o compiuto atti tipici del mandato parlamentare su questa vicenda per la bellezza di trentotto Il fatto che sulla stessa questione il senatore Albertini si sia esposto anche durante la XVII legislatura nazionale, cioè quella in essere, non può essere ritenuto irrilevante. Anzi, è proprio questo il presupposto per radicare la competenza della Giunta prima e dell'Assemblea dopo. Le ulteriori esternazioni contestate al senatore Albertini in pendenza del mandato di parlamentare italiano sono infatti state numerosissime e pienamente coincidenti in termini di oggetto, materia, presupposti, fatti Grazie, Invece, si è in presenza di quella naturale prosecuzione dell'attività di manifestazione del pensiero e di critica di politica giudiziaria che è propria dell'esercizio del mandato parlamentare; essa si pone in diretta connessione teleologica con le prime esternazioni (esposto del 22 ottobre 2012),

credo che tutti i colleghi siano in grado di scoprirlo da soli. Rileva chiarire che, in termini di imputazione penale, la calunnia aggravata che si contestava all'allora parlamentare europeo Gabriele Albertini è stata reiterata, ribadita, meglio precisata. tutto evidente che la continuità assoluta dell'operato del senatore pretenderebbe uno scrutinio dei profili di insindacabilità fondati sulla continuità e la coerenza logica delle sue condotte. In questo senso, peraltro, il fatto che il Parlamento europeo abbia declinato la guarentigia dell'insindacabilità non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di un nesso diretto ed evidente tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari è argomento in più perché l'Assemblea si pronunci nel merito del *fumus persecutionis* e riconosca la piena sussistenza del nesso funzionale delle dichiarazioni del senatore rese *extramoenia* con una condotta da parlamentare perfettamente conseguente. Ma vi è ancora di più. Vale la pena notare che lo stesso protocollo n. 7 per i privilegi e le immunità dell'Unione europea impone che: «Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Paese». Nel caso di specie si realizzerebbe proprio l'inverso, cioè trascurando il legame di tutta evidenza e, dalla prospettiva dell'incriminazione penale, il vincolo di continuazione che congiunge tutte le condotte del senatore*...

sostanzialmente il senatore in una zona grigia di mancata protezione, derivante dalla teorica estensione del principio restrittivo dell'insindacabilità parlamentare europea. Tutto ciò in danno della latitudine applicativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione italiana. Tralascio il commento delle sentenze già citate proprio alla luce di tali conclusioni, si prospetta la necessità che l'Assemblea del Senato si dichiari competente a valutare nel merito il nesso funzionale tra le dichiarazioni di Gabriele Albertini e la sua carica di senatore, alla luce dell'intera vicenda che lo ha visto opporsi all'agire del visto opporsi all'agire del magistrato requirente, che è parte nel processo penale a suo carico. È inoltre necessario che l'Assemblea consideri le plurime dichiarazioni rese dal senatore Albertini, ivi comprese quelle contenute nell'esposto del 22 ottobre 2012, coperte dalla scriminante di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, perché in connessione logica e funzionale fra di loro. Da ciò discende l'esclusione dell'antigiuridicità delle dichiarazioni per le quali il senatore Albertini è gravato dell'addebito di calunnia aggravata. Per tali motivi, la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Albertini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

di segnalare le sentenze della Corte di cassazione del 2004 e del 2007,

tralasciò quest'Assemblea del Senato quando il 14 dicembre 2014 affermò la propria incompetenza devolvendo al Parlamento europeo la decisione sul punto. va segnalato il tentativo sterile, incapace di approfondire i temi sottesi alla questione, vale a dire il reato continuato di cui all'articolo 81 del codice penale e l'articolo 16 che radica la competenza quando vi è un'ipotesi di reato continuato. Tutto questo oggi, in una relazione

senatore Albertini. Tuttavia, se mi consente, vi giungo con un ragionamento tecnicamente più corretto; un ragionamento tecnico

tralasciano l'esame delle dichiarazioni di Albertini che andavano in una direzione che vi dirò di qui a poco in sede di dichiarazione di voto, e non nella direzione che loro avevano individuato la prima volta, il 14 dicembre del 2014.

che sbagliavate nel 2014. Oggi non si può giungere alla conclusione alla quale giungemmo noi nel 2014 - e giungiamo oggi in questa Assemblea - con un sorvolamento di argomenti che forse in quel momento erano Il Partito Democratico è a corrente alternata; io non so quali ragioni oggi inducano questa questa maggioranza a giungere a una conclusione diametralmente opposta a quella di alcuni mesi fa. Per la verità, posso immaginarle perché a me non manca l'immaginazione, però non mi lascio trascinare da quella cultura dell'opposizione «comunque e ad ogni costo». Sono felice che siate giunti alla conclusione a cui siete giunti; sono felice per voi perché in questo modo cominciate a dare segnali - che secondo me dovreste dare in maniera più forte, più decisa, più determinata - di garantismo e di tutela delle nostre funzioni e delle istituzioni del nostro Paese.

proprio in tema di corretta applicazione dell'articolo 16 del codice di procedura penale, dell'articolo 81 del codice penale e dell'interpretazione delle sentenze della Corte di cassazione (ben due) del 2004 e del 2007 in tema di indagine indagine relativa alla corretta applicazione del citato Protocollo n. 7, in particolare dell'ex articolo 10, oggi articolo 9. Dopo ve lo dirò.

quando nell'ambito di questa procedura il primo relatore nominato dal Presidente della Giunta delle immunità illustrò le sue considerazioni e conclusioni durante la seduta del 24 novembre del 2015 chiedendo il sostanziale rigetto della pretesa del senatore Albertini, mi ritrovai nelle sue lineari e trasparenti richieste giuridicamente e politicamente, anche perché confermavano la precedente decisione della Giunta delle immunità e dell'Aula del Senato in relazione alla causa civile per la quale, parimenti, il senatore Albertini aveva richiesto e pretendeva l'immunità, che correttamente, correttamente, relativamente alla causa civile, Giunta e Senato avevano negato. Quando, però, nella seduta del 5 ottobre 2016 il nuovo relatore, nominato a seguito di rinunzia del primo, modificò totalmente le precedenti conclusioni,

mi resi conto che molto non quadrava e cominciai in Giunta a chiedere di conoscere il capo di imputazione, che allora sembrava non risultare nemmeno alla seconda relatrice nella sua esatta configurazione. Inopinatamente, la Giunta decise a maggioranza di non acquisire nemmeno la richiesta di rinvio a giudizio, dalla quale si sarebbe potuto desumere con precisione il capo di accusa. Comunque, dalle pieghe e dai risvolti del fascicolo, siamo riusciti a individuare il capo di imputazione e a sapere, quindi, che il tribunale sta procedendo nei confronti del senatore Albertini per fatti commessi fino all'ottobre del 2012, quando cioè il dottor Gabriele Albertini non era nemmeno senatore. Ricordo che il capo di imputazione viene fissato non certo dalla Giunta o dalla relatrice e non certo dal Senato. Nemmeno il tribunale lo può cambiare d'ufficio o d'autorità. Il capo di imputazione viene fissato all'inizio per principio costituzionale e su quello bisogna decidere. Quindi, il capo di imputazione fa riferimento all'ottobre del 2012. Il dottor Albertini non era senatore e, quindi, la questione dovrebbe semplicemente finire qui, senza dover andare a discutere di articolo 81, che non è nemmeno contestato nel capo di imputazione o di date diverse e successive. La richiesta odierna della relatrice però mi costringe

«I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Questo è il principio che va applicato. Il secondo comma fa riferimento fa riferimento a tutt'altra fattispecie e, cioè, a quella di interventi di natura cautelare, reale o personale, come il provvedimento restrittivo, come le perquisizioni, come i sequestri, per i quali ci vuole l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene. Nel momento in cui viene richiesto il provvedimento, va valutato se la persona fa parte di un ramo del Parlamento. Tutt'altra situazione, come ricordavo e leggevo, è quella che fa riferimento al primo comma, secondo cui i voti e le opinioni devono fare riferimento all'esercizio delle funzioni. funzioni. Il principio costituzionale è chiarissimo. Ricordo un brocardo latino: *in claris non fit interpretatio*. Non si tratta di discutere dei rapporti tra il dottor Robledo e l'attuale senatore Albertini, degli scontri e delle polemiche, anche piuttosto dure, che ci sono state. Ci sono settori e ambiti diversi che ne stanno discutendo; c'è una causa civile pendente: c'è un procedimento penale, come abbiamo saputo poco fa; c'è stato un procedimento sostanzialmente disciplinare di trasferimento del dottor Robledo da parte del Consiglio superiore della magistratura. Questi sono però gli ambiti istituzionalmente corretti per intervenire su tali vicende.

Dico questo perché nella lunga arrampicata sugli specchi si cerca di rinvenire e utilizzare criteri ermeneutici della suprema Corte di cassazione per dirimere tutta la questione. Tra l'altro, almeno a mio parere, la suprema Corte di cassazione è citata

da una parte sostanziali e dall'altra procedurali, per l'applicazione di questo privilegio o immunità ai parlamentari europei, così come ai parlamentari italiani. Ho detto che basta leggere perché non bisogna fermarsi alla prima parte, che magari in qualche situazione può far comodo, ma bisogna leggerla fino in fondo, perché si tratta anzitutto di un riferimento al Protocollo Europeo in questione citato anche dal regolamento europeo del 2014. L'articolo 9 del Protocollo stabilisce,

a motivo delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Questa norma del Parlamento europeo è chiarissima. Anche quando si fa riferimento a tutte le altre norme successive del Parlamento europeo

che l'articolo 9 del regolamento fa riferimento alle procedure in materia di immunità per i parlamentari europei. Ciò vuol dire che se nella sostanza si applica il concetto di immunità vigente nello Stato da cui proviene il parlamentare europeo, per quanto riguarda le procedure vanno seguite

sia stata presentata una richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituiscano, tra le altre cose, un ostacolo all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del mandato. Questa è la sostanza e la procedura viene espressamente indicata: Commissione, *plenum*, possibilità di revoca. Leggiamo quindi fino in fondo queste norme e distinguiamo la tutela sostanziale dalle linee procedurali. Concludo rapidamente il mio intervento dicendo che non siamo tenuti e non dobbiamo intervenire sui rapporti tra due persone. Noi dobbiamo ragionare in materia costituzionale, senza far riferimento a dichiarazioni rese nell'attività di sindaco e, poi, di europarlamentare. Si tratta di giudicare se, nell'esercizio delle funzioni di senatore, si è verificata la situazione così come contestata. Quindi per questo, a mio modo vedere, in prima battuta non saremmo nemmeno competenti,

per sostenere che le dichiarazioni in questione siano state rese nell'esercizio delle funzioni di senatore. Signora Presidente, tralascio di intervenire sui presupposti dell'insindacabilità perché la relazione costituisce un documento fin troppo sufficiente al fine di dimostrare che le dichiarazioni del senatore Albertini siano state rese sotto l'ombrello della copertura costituito dall'articolo 68 della nostra Costituzione. Intervengo piuttosto sul problema della competenza perché lo stimo oggetto di fraintendimenti e soprattutto perché costituisce l'aspetto preliminare È chiaro che noi possiamo interessarci della sindacabilità o meno una volta che si sia stabilito che il Parlamento italiano è competente a valutare le dichiarazioni del senatore Albertini. Orbene, il fraintendimento riguarda proprio l'aspetto della competenza perché omette di valutare non soltanto l'articolo 3 del Regolamento del Parlamento europeo ma anche l'articolo 9 del protocollo n. 34 delle guarentigie e delle immunità il cui testo, al contrario di ciò che ho sentito più volte dire in contesti che sono sempre stati obiettati anche nel corso dei lavori della Giunta delle elezioni delle elezioni e delle immunità parlamentari, nelle sue doppie lettere *a)* e *b)* è assolutamente chiaro nell'affermare un principio che ci si ostina a non comprendere. Il principio è il seguente e la lettura del testo darà conferma della bontà delle mie modeste convinzioni, che d'altronde sono perfettamente corrispondenti a quello che ben due sentenze della Corte di cassazione, dedicate espressamente all'argomento, hanno in maniera assolutamente concorde affermato. L'articolo 9 contiene una sorta di clausola dell'equivalenza. Si dice sostanzialmente alla lettera *a)* che il parlamentare europeo per i fatti commessi nel territorio dello Stato di appartenenza soggiace alle guarentigie e ai criteri di tutela stabiliti dall'ordinamento interno di appartenenza. La norma è chiarissima nella sua formulazione letterale. il testo stabilisce un principio diverso secondo il quale il parlamentare europeo è, al contrario, assoggettato a diversa disciplina tutte le volte in cui il fatto sia stato commesso all'interno dei territori di Stati membri diversi, ovviamente, dallo Stato di appartenenza originaria del parlamentare. noi non possiamo sfuggire a questa distribuzione della competenza che si regge su una regola storica per ogni tipo di procedimento, quella cioè costituita

come stabilisce la Corte di cassazione, un rinvio perfettamente ricettizio della disciplina nazionale di guarentigia ai fatti commessi in territorio italiano dal parlamentare europeo, sicché noi abbiamo una situazione assolutamente chiara: il parlamentare italiano che abbia commesso in territorio italiano un fatto che si stima stima si debba valutare alla stregua del primo comma dell'articolo 68, soggiace a questa disciplina. Pertanto, e lo dico con assoluta certezza morale, è perfettamente irrilevante citare l'articolo 68 nella sua articolazione, ossia laddove si parla di esercizio delle funzioni. l'esercizio delle funzioni di parlamentare europeo è perfettamente equivalente all'esercizio delle funzioni di parlamentare nazionale

che determina questa perfetta sovrapposizione, nel senso che al parlamentare europeo - lo dico per l'ennesima volta - si applica la disciplina giuridica che si applica a un parlamentare nazionale. Vi è di più e questo lo dice chiaramente la Corte di cassazione: non si applica solo la disciplina di diritto sostanziale, ossia la disciplina giuridica delle immunità,

di tutte le fasi procedimentali anche nell'individuazione degli organi preposti all'applicazione dell'articolo 68 e all'affermazione della sussistenza dei suoi presupposti. Questa affermazione - ripeto - non sta soltanto nella buona lettura del testo dell'articolo 9 del protocollo, che è la norma di collegamento tra la qualifica di parlamentare europeo e la sottomissione alla disciplina dell'articolo 68,

sottoposti alla valutazione della Corte di cassazione si trattava di affermare se il parlamentare europeo dovesse godere della maggiore e più ampia disciplina fissata dalle regole europee, cioè dal protocollo n. 34, ovvero dalla ben più limitata guarentigia fissata dell'articolo 68 della nostra Costituzione. 10, ora 9, del protocollo sui privilegi e sulle immunità stabilisce non soltanto che il parlamentare europeo non può essere detenuto, ma addirittura stabilisce che non può essere sottoposto ad alcuna forma di procedimento giudiziario. La Corte di cassazione, nel decidere questa distribuzione della competenza, escluse che un parlamentare italiano potesse giovarsi della ben più favorevole disciplina dell'articolo 10, ora articolo 9,

dei quali ci stiamo occupando, ma anche la giurisprudenza richiamata nella relazione della senatrice Filippin per giungere alle conclusioni che mi permetto soltanto di suggerire all'Assemblea, vorrei indicare un'ulteriore circostanza. Il senatore Albertini concretizza nella sua figura una sorta di duplice funzione:

quello degli effetti di un eventuale giudizio, perché l'organo politico pregiudicato da un eventuale procedimento penale che sfociasse in una sentenza sarebbe, per l'appunto, il Senato della Repubblica. non soltanto vale la regola in virtù della quale il parlamentare europeo, se commette un fatto sul territorio nazionale, come sarebbe avvenuto nel caso di Albertini, soggiace, in virtù dell'articolo 9, norma interposta per effetto delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale, ma appartiene a quell'organo, Senato della Repubblica, che subirebbe gli effetti di una sentenza pronunciata nei suoi confronti.

non può comportare che non si debbano applicare i principi stabiliti da quelle sentenze richiamate sia dalla relatrice (sono contenuti nella per sgombrare definitivamente il campo da qualsiasi equivoco. Qui dobbiamo cercare di comprendere ciò che il senatore Albertini ha posto in essere e che che è ben spiegato nella relazione, che vi invito a leggere; purtroppo il tempo è stato tiranno e non è stato possibile alla relatrice far conoscere gli esatti contorni di tutta la vicenda. Ma, leggendo la relazione depositata agli atti, si comprende cosa sia accaduto in questa vicenda. È pur vero, come ha già spiegato il senatore

Dicevo quindi che quella serie di comportamenti, che si sono reiterati per ben trentotto volte e che hanno originato trentotto procedimenti, non possono essere considerati singolarmente, ma vanno valutati nella loro complessità e nella loro interezza, uniti - come è ben spiegato nella relazione - sotto il cosiddetto vincolo della continuazione, previsto dall'articolo 81 del codice penale. È detto anche - voglio leggere questa parte della relazione - che, ove si ragionasse in maniera differente, cioè se

si sarebbe trovato e si troverebbe sprovvisto di qualsiasi tutela, pur essendo acclarato - credo che anche le pronunce del Consiglio superiore della magistratura, richiamate dalla relatrice nella lettura della sua relazione, confermino in maniera innegabile - che c'era stato un atteggiamento che possiamo sicuramente considerare come persecutorio nei confronti del senatore Albertini. Ciò ha indotto quindi la Giunta ad assumere la decisione che è stata assunta, senza modificare i suoi orientamenti. Voglio anche ricordare che la prima decisione era stata assunta era stata assunta sulla base di un solo fatto; ma la domanda che è stata proposta dal senatore Albertini nella vicenda della quale oggi ci stiamo occupando, e che ha indotto la Giunta ad assumere la decisione di formulare la proposta di insindacabilità, riguarda invece l'interezza dei suoi comportamenti. Di questo stiamo parlando. Stiamo valutando, come dobbiamo sempre fare nell'adottare le nostre decisioni, se ci sia stato un atteggiamento persecutorio nei confronti del parlamentare. Abbiamo accertato, abbiamo appurato e ci siamo convinti che questo atteggiamento persecutorio ci sia stato; in questo senso, quindi, è stata avanzata Di questo stiamo parlando. C'è poi la giurisprudenza della Corte costituzionale, mirabilmente e magistralmente richiamata dal collega D'Ascola, che sgombra il campo da qualsiasi equivoco, anche sotto il profilo del diritto. mi pare che la vicenda possa considerarsi assolutamente definita nei suoi contorni e che la decisione assunta sia assolutamente quella

Voglio soltanto accennare ad alcuni argomenti per sgombrare il campo da alcuni equivoci che hanno indotto a valutazioni del tutto fuorvianti. I motivi di dissapore tra me e il dottor Robledo sono noti e vengono da lontano. Egli cercò in ogni modo di far emergere addebiti penalmente rilevanti negli anni in cui io vestivo i panni di sindaco della città di Milano. Nulla da obiettare da parte mia, salvo difendermi; evidentemente, egli aveva le sue ragioni per ritenermi meritevole di tanta attenzione. Come tutti sappiamo, il pubblico ministero ha il diritto e il dovere di esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione. Tuttavia, una volta dismessi i panni di sindaco ed eletto al Parlamento europeo, ritenni di difendermi in pubblico da queste sue attenzioni, che io so essere indebite e soprattutto esercitate con metodi indegni delle funzioni giudiziarie in una moderna democrazia avanzata. Fu allora che mi espressi, in alcune interviste, in termini assai critici sui metodi impiegati dal dottor Robledo nello svolgere le proprie funzioni requirenti e, precisamente, pronunciai le parole «metodi da Gestapo», riferendomi in particolare al modo in cui vennero trattate alcune persone, informate dei fatti, nel corso delle indagini condotte dallo stesso dottor Robledo. Venni querelato per diffamazione. Ricevuta la citazione, e nel corso del tentativo obbligatorio di mediazione, mi offrii persino di raggiungere un accordo che potesse chiudere la disputa (beninteso, senza alcuna ritrattazione delle critiche) chiedendo però che l'ammontare di denaro da me offerto (35.000 euro) venisse devoluto in beneficienza all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri o ad altra ONG a scelta dell'attore, per un fine nobile. Il dottor Robledo ricusò l'offerta e da ciò compresi che egli intendeva ottenere una somma di denaro da tenere per sé, ritenendo che potesse cancellare la terribile macchia costituita dalle mie parole. Conclusosi il processo, la sentenza civile, lo scorso 2 settembre, tra l'altro, così si esprime sul punto: «Correttamente sono stati evidenziati, dalla difesa convenuta, gli elementi conosciuti e conoscibili dal senatore Albertini al momento in cui rese le sue dichiarazioni alla stampa, affermando che da parte del pubblico assegnatario del procedimento fossero stati usati comportamenti definibili come «metodi da Gestapo». Orbene, detti elementi erano costituiti dalle dichiarazioni che Giancarlo Penco aveva personalmente reso all'allora sindaco di Milano Albertini, alla presenza di più persone». Vi risparmio la lettura di tutti questo argomenti, che però lascerò per la

quantomeno "putativa", del passo: «l'inchiesta parte dallo stesso pubblico ministero che interrogava di notte con metodi da Gestapo i consiglieri comunali (…)». Emerge, inoltre, anche la verità fattuale.

la sottoscrizione di emendamenti in bianco al Consiglio comunale. Gli stessi argomenti delle interviste furono oggetto di un esposto al Ministro della giustizia. Ne seguì la denuncia per calunnia aggravata di cui stiamo parlando ora.

Il procedimento condotto presso quella Assemblea si concluse con esito negativo. Con mia grande sorpresa, l'Assemblea rappresentativa europea non ritenne di considerare le mie dichiarazioni coperte dal raggio di azione dell'immunità derivante dalla carica elettiva. È già stato ricordato il perché ciò è sorprendente. Tuttavia - e questo è il punto - la spiegazione di questo esito doveva venire alla luce nei mesi successivi al voto di Bruxelles, quando venni a sapere che il dottor Robledo si era adoperato per incidere sull'istruttoria relativa all'insindacabilità delle opinioni da me espresse, e aveva posto in essere una condotta stigmatizzabile. Già come parte di un processo tra privati - quello in cui egli era parte offesa denunziante per calunnia aggravata - avrebbe dovuto esimersi da qualunque intervento nelle sedi precipue in cui gli organi parlamentari, e solo essi, debbono poter valutare la fondatezza della richiesta di attivazione della prerogativa. Ma ciò egli avrebbe dovuto fare a maggior ragione come magistrato della Repubblica, il quale non dovrebbe tendere ad influenzare, in un modo o nell'altro, lo svolgimento di un potere proprio di un altro potere (nel caso, persino sovranazionale e avvalendosi di collegamenti e aderenze improprie e ambigue). Questo non sono certo io ad affermarlo, il che potrebbe apparire un argomento in certa misura partigiano o fazioso. Questa volta tutto assume una luce obiettiva, certa e al momento il dottor Robledo ha subito una condanna da parte della sezione disciplinare del CSM che, dopo avergli inflitto una sanzione in sede provvisoria e cautelare, ha poi confermato la fondatezza dell'addebito e dell'incolpazione, condannandolo anche nel merito pieno e disponendone il trasferimento da Milano a Torino. Il dispositivo pubblicato dalla sezione disciplinare del CSM lo scorso 11 novembre dichiara colpevole il dottor Robledo proprio nel capo d'incolpazione relativo alle sue indebite interferenze per influenzare e modificare il corso e l'esito del procedimento del Parlamento europeo che mi riguardava. caso, nel resoconto stenografico troverete tutti gli elementi di tali disposizioni, con il Capo I e II del dispositivo della sezione disciplinare che riguarda proprio le azioni che sono state perpetrate dal dottor Robledo divulgando notizie inerenti a indagini in corso effettuate dal suo ufficio e ricevendo in cambio informazioni riguardanti il mio procedimento per far arrivare - come di fatto avvenne - una contromemoria. Sottolineo che sino ad ora ho mantenuto la descrizione degli eventi su un tono volutamente asettico, senza esprimere giudizi di sorta se non sulla scorta delle pronunce di un organo giurisdizionale qual è la sezione disciplinare del Ma vi è di più. Quando, lo scorso 3 novembre, sembrava che questa Assemblea dovesse procedere al voto sulla proposta deliberata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità il 25 ottobre il dottor Robledo si spingeva oltre. Con un comunicato denominato «petizione» si prodigava in una raccolta di firme contro quella ormai prossima delibera del Senato che egli si permetteva di qualificare come prova di un «privilegio insopportabile»; e quale effetto od oggetto od oggetto di un «voto di scambio ignobile». Rivolgeva poi altri epiteti a questa Assemblea e concludeva con il diffamarmi dando credito all'idea secondo cui io avrei minacciato di revocare il mio supporto al Governo se non mi si fosse concessa l'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

hanno sottoscritto un'interrogazione (faccio osservare che sono uno in più dell'ultima fiducia al Governo Renzi e cinque in più della prima fiducia al Governo Gentiloni), in cui si chiede al Ministro della giustizia di avviare l'azione disciplinare nei riguardi di tale magistrato.

è la difesa dell'indipendenza del Parlamento e della distinzione dei poteri che fa capo al fondamento della nostra libertà e della nostra Repubblica. *(Applausi dai Gruppi*

inducono il nostro Gruppo a ritenere l'insindacabilità delle condotte del senatore Albertini. c'è chi in quest'Aula non riesce a spogliarsi delle vesti di magistrato, di giudicante, per indossare quelle del parlamentare.

a spogliarsi della sua cultura di magistrato per assumere, condividere e sposare quella di membro

modo dobbiamo dire che c'è un concorso di reati che muovono dal 2012 per arrivare al 2016, per cui la competenza, in mancanza di una maggiore gravità però, caro senatore Casson, stiamo facendo una causa. causa. Stiamo trasformando l'Aula del Senato in un'aula giudiziaria e questo non è consentito, non è corretto. Noi qui dobbiamo adempiere ad una funzione che il popolo italiano ci ha assegnato, ben diversa rispetto a quella che viene conferita al magistrato che supera il concorso in magistratura. Noi dobbiamo guardare la vicenda nella sua univocità. Non possiamo trascurare il fatto che le condotte del senatore Albertini vanno viste, analizzate e approfondite nella loro complessità, senza procedere ad un'applicazione rigorosa della norma. Che cosa ha fatto il senatore Albertini? Questo è quello che dobbiamo valutare in quest'Aula; questo è quello che la maggioranza non è riuscita a fare in altri casi. venga, quindi, se quest'oggi, almeno per la vicenda del senatore Albertini, si riesce a ragionare in maniera corretta. Cosa ha fatto il senatore Albertini, ha forse difeso se stesso? Direi di no. ha tutelato un organismo istituzionale del nostro Paese, vale a dire il Consiglio comunale di una delle più importanti città italiane. Le attività di indagine non erano dirette esclusivamente sul sindaco di allora, senatore Albertini, ma andavano a colpire il Consiglio comunale di Milano e il senatore Albertini, ancorché non fosse più sindaco di quella città ma europarlamentare, ha inteso

sostanza, il senatore Albertini ha esercitato un potere che gli era proprio in quanto europarlamentare e in quanto oggi parlamentare del nostro Paese; un potere di controllo

ha inteso denunciare un qualcosa che comprometteva in maniera seria l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Vedete, colleghi,

in nome del popolo italiano, dobbiamo innanzitutto tutelare. Il senatore Albertini ha invocato il rispetto di questo equilibrio tra i poteri dello Stato e lo ha fatto in una prospettiva che va al di là della sua difesa personale, perché non stava difendendo sé stesso da un'accusa che veniva mossa a lui nell'esercizio della funzione di sindaco; la sua difesa andava al di là, andava a tutelare l'intero Consiglio comunale di Milano rispetto a delle condotte di un magistrato che,

come e per cosa un rappresentante del Parlamento viene accusato, indagato, perquisito, o ahimè arrestato. Questo è un nostro dovere. la maggioranza, con questa relazione della senatrice Filippin, prende una decisione che va nella giusta

per una serie di ragioni e anche di disattenzioni da parte dell'organizzazione di questa Camera del Parlamento italiano.

avremmo potuto dare un contributo di garantismo anche nelle sedi istituzionali più ristrette come la Giunta, ma non ci è stato consentito. Forse la nostra cultura garantista e liberale in un certo senso spaventa chi ritiene di voler rimanere arroccato su quella giustizialista. si dà un segnale flebile, ne prendiamo atto. Lo condividiamo, esprimiamo anche apprezzamento e diciamo: di tanto in tanto, imparate anche ad ascoltare voci liberali che possono darvi suggerimenti che vanno nella direzione dell'affermazione della democrazia nel nostro Paese e, in questo caso specifico, nel rispetto di quell'equilibrio tra tra i poteri dello Stato che, come vi ho detto, è un elemento portante della democrazia di un gruppo sociale e di un popolo. Signora Presidente, colleghi, il mio intervento, come è ovvio su queste materie, sarà a titolo personale, come sempre è a titolo personale all'interno della Giunta che ha segnalato in via preliminare la questione. infatti che, nel momento in cui dobbiamo giudicare certe situazioni, non possiamo affidarci alla collegialità di Gruppo ma fare i conti direttamente con la nostra coscienza e con i dati di conoscenza che abbiamo avuto a disposizione. Per quanto riguarda gli elementi tecnici - mi riferisco alla mirabile e coraggiosa relazione della collega, senatrice Filippin, e del presidente della Commissione giustizia del Senato, senatore D'Ascola le questioni dal punto di vista giuridico sono quelle; i fatti sono quelli. Vi è, però, una questione, colleghi, sulla quale credo che dobbiamo soffermarci, ed è la questione delle questioni, che questa esperienza del collega Albertini mette in risalto in maniera inequivocabile: nella nostra attività di parlamentari europei, italiani, senatori e deputati, possiamo permetterci di criticare e di richiamare l'attenzione di quanti hanno il dovere di vigilare sul comportamento degli intoccabili? Questa è la questione. Ed è la questione che si trascina ormai da decenni, colleghi, perché viviamo in un sistema squilibrato, in un sistema in cui siamo siamo sottoposti a giudizio, noi investiti dalla sovranità popolare; altri, invece, sottopongono a giudizio altre istituzioni e soggetti pubblici e privati senza rispondere ad alcuno, se non al loro organo di autogoverno, che spesso - mi permetto di dire - ha la sordina. la sordina. Riconosco all'attuale Consiglio superiore della magistratura un certo attivismo, anche nella direzione di una verifica dei comportamenti dei propri autogovernati, però ci vuole più coraggio, ci vuole più tempistica; non si può arrivare alle vicende milanesi di uno scontro esplicito, diretto e quotidiano tra operatori della giustizia senza che vi siano gli interventi necessari. Questa vicenda, collega Albertini, arriva da quel mondo lì, nel momento in cui il collega Albertini ha avuto il coraggio di porre la questione delle questioni. che allora, colleghi, questo non è un problema solo di tecnicalità giuridica; è un problema del nostro agire politico: possiamo esercitare fino in fondo la nostra funzione di legislatori e anche di ispettori, con le nostre prerogative parlamentari, nei confronti di altri oppure no? Se oggi il responso nei confronti della relazione della Giunta fosse negativo, chi si sente di presentare un atto di sindacato ispettivo verso quegli ambienti?

muoversi nella legittimità della sua condizione di difendersi da un'accusa che ritiene infamante (l'avere usato metodi da Gestapo: quanti metodi da Gestapo, collega Albertini, abbiamo dovuto patire e subire in questi decenni nel nostro Paese?), ma si permette anche di intervenire sull'attività di organi costituzionali.

della Corte di cassazione (non solo una, per la verità) che spesso dimentichiamo quando dobbiamo fregare qualcun altro. Lo dico anche in funzione della Giunta perché, non sempre, come nel caso del collega Albertini la prima volta, il richiamo a questa competenza, che era già evidenziata nelle sentenze della Corte del 2004 e negli anni successivi; Senato italiano, in questo caso specifico, a giudicare secondo la normativa vigente in Italia un parlamentare, allora europeo e ora italiano, che eventualmente ha commesso un reato nel territorio italiano.

un fallo fuori area non è rigore. Mi pare che questa cosa la capiscano anche i bambini che si approcciano al calcio. Un fallo fuori area non sarà mai rigore, anche se continua dentro l'area di rigore. Se inizia fuori area; è fuori area. Questo lo porto come esempio per capire di cosa stiamo parlando. Il senatore Albertini ha commesso un reato; lo ha detto adesso il collega Buemi. Ha parlato di reato. *(Commenti del senatore

Dopodiché viene eletto senatore e poiché è eletto parlamentare interviene una specie di amnistia di tutti i reati precedentemente commessi qualora li reitera

Allora a questo punto mi rivolgo ai colleghi: se avete fatto delle calunnie prima di entrare in Parlamento, reiteratele ora, perché, continuando, facciamo un bel *link* e diciamo che il reato è continuato e questo e quello che avete fatto prima viene assolto

al Parlamento europeo, che gli ha detto: no, non esiste alcun nesso funzionale tra la tua attività politica e ciò che ha dichiarato. Il senatore Albertini ha chiesto al Parlamento europeo di riesaminare la sua istanza, e il Parlamento europeo gli ha detto: allora non hai capito bene, ti abbiamo già detto che non c'è nesso funzionale, basta, smettila. E per la seconda volta ha

«Evidenzio preliminarmente che l'articolo 68, comma 1, della Costituzione costituisce una garanzia funzionale all'esercizio dell'attività parlamentare e non può configurarsi quindi come un privilegio. Di conseguenza, tale prerogativa non può essere applicata al di fuori del contesto di riferimento, dovendo essere specificatamente correlata all'espressione di opinioni legate da un nesso funzionale con l'attività parlamentare». reiterato quanto era già stato detto prima. Ebbene, a un certo punto succede qualcosa di strano. Questi sono i fatti, che qui espongo: arrivano alcune dichiarazioni

la richiesta di rinviare la discussione e la votazione sulla proposta del senatore Pagliari di rigettare la richiesta del senatore Albertini.

dal ruolo di relatore. Si sente offeso, probabilmente in un rigurgito di orgoglio di persona che conosce un po' il diritto si di cosa stiamo parlando? Cosa mi state facendo fare? Cosa mi volete obbligare a fare? Questa stessa faccia la vedo oggi anche nel senatore Cucca e in tutti i colleghi

in Giunta, in particolare dal senatore Caliendo e dal senatore Alicata, e a quanto è stato detto in quest'Aula dalla relatrice Filippin e dal presidente D'Ascola e non mi dilungo sulle argomentazioni

le precise ragioni giuridiche che sono state citate, le tutele, a nostro parere, gli sono dovute. Vorrei anche aggiungere un altro elemento che non è stato menzionato. Ci stiamo occupando di una vicenda

Le ha espresse non per difendere se stesso da una qualche accusa che gli era stata rivolta, perché nessuna accusa gli era stata rivolta, ma per difendere l'interesse pubblico nella vicenda alle azioni della Milano - Serravalle, dove la Corte dei conti ha accertato un danno erariale di 118 milioni di euro. Gabriele Albertini,

Bisognerebbe capire perché il senatore Albertini ha espresso quelle parole: lo ha fatto a difesa dell'interesse pubblico, perché si trovassero i colpevoli un ammanco, di un danno erariale di 118 milioni di euro. Credo che questo, anche agli elettori del Movimento 5 Stelle, interessi di più che non la singola situazione del senatore Albertini oggi. Pertanto questo è il quadro: il senatore Albertini non se l'è presa improvvisamente Questo magistrato ha presentato denuncia per calunnia a seguito delle parole di Gabriele Albertini, che ha lamentato la scarsa efficacia di queste indagini. Non entriamo nel merito perché non è questo il punto, questa è l'origine della vicenda. Noi, come

ci siamo espressi per la insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Albertini. Ci esprimiamo allo stesso modo oggi. Rileviamo che nella fase precedente, quando ci si riferiva all'azione civilistica, il responso di questa Assemblea non fu favorevole al senatore Albertini e apprezziamo che si sia assunta una posizione diversa. Sarebbe interessante analizzare le cause e forse, più che le cause, i tempi in cui sono stati

ci sono tutte le premesse per ritenere che le parole per le quali è stato accusato il senatore Albertini debbano essere coperte dall'insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione, non a difesa della singola persona, in questo caso non a difesa di Gabriele Albertini, ma a difesa della facoltà di un parlamentare di perseguire l'interesse pubblico (e direi che in questo caso è particolarmente evidente che si perseguiva l'interesse pubblico), anche in un modo aspro che in altre circostanze potrebbe essere eventualmente perseguito. Naturalmente si potrebbe entrare nel merito, ma non è questa la sede.

nel Gruppo di Forza Italia. L'indicazione per il Gruppo di Forza Italia è quello della libertà di voto e dunque un richiamo alla coscienza di ogni senatore del nostro Gruppo, di valutare

in una decisione di questo genere, che non è una decisione politica. Se fosse una questione politica potremmo metterla sul piano della maggioranza e dell'opposizione, per cui il senatore Albertini fa parte della maggioranza e noi siamo all'opposizione, ma non abbiamo applicato questa dinamica in alcun caso, né quando si trattava di persona della nostra stessa parte politica, né quando si trattava di avversario politico e non l'applichiamo oggi. Ci appelliamo alla coscienza di ciascuno e ci auguriamo che tutti lo facciano,

in ogni altra occasione analoga.

il senatore Albertini è un uomo d'onore e una persona che abbiamo apprezzato molte volte per i suoi interventi. Tuttavia, non possiamo votare a favore di maggioranza, perché con tutta evidenza i fatti si riferiscono a un periodo in cui il senatore Albertini non era senatore e perché il Parlamento europeo, dal nostro punto di vista, istituzionale, non sindacabile, per tre volte ha ritenuto di non poter dare ragione alle richieste del senatore Albertini e sarebbe del tutto improprio che il Senato decidesse oggi

possono apparire in molti passaggi diversificate e in parte contrastanti. La cosa non stupisce ed è in parte legata alla delicata valutazione di una vicenda che è stata al centro di polemiche pubbliche anche aspre, soprattutto in considerazione dell'eccezionalità della circostanza, data dal fatto che le opinioni del senatore Albertini oggetto di censura sono state espresse «non solo in pendenza del mandato di parlamentare italiano», ma anche nel periodo in cui egli era sindaco di Milano ed europarlamentare. Grazie, Presidente. Se infatti, di per sé, da un lato si afferma che il requisito minimo per far valere la guarentigia dell'insindacabilità è quello che il parlamentare sia in carica nel momento in cui si svolge il fatto di cui si contesta la liceità, tuttavia - ci è stato ricordato - le dichiarazioni del senatore Albertini possono anche essere contestualizzate in un quadro ben più ampio, come denota il fatto che lo stesso Albertini abbia svolto interventi collegati o compiuto atti tipici del mandato parlamentare per ben trentotto volte, anche nel corso della presente legislatura. Credo allora che proprio tale situazione, indubbiamente *sui generis*, possa spiegare meglio di ogni polemica le posizioni emerse durante i lavori della Giunta, alcune volte a negare la sussistenza del nesso funzionale e quindi della prerogativa dell'insindacabilità, altre invece di segno diametralmente opposto, le quali hanno poi finito per prevalere in seno al Collegio. Senza entrare ulteriormente nella questione, va ribadito dunque che oggi l'Assemblea del Senato è chiamata a pronunciarsi non sulle eventuali responsabilità penali del senatore Albertini, ma esclusivamente sulla sussistenza o meno del nesso funzionale sull'applicabilità o meno della garanzia parlamentare dell'insindacabilità. Tale valutazione, come è evidente, è estremamente delicata e articolata e ogni singolo senatore sarà chiamato ad esaminare con attenzione la decisione assunta dalla Giunta nel caso in esame, valutandone la scelta di considerare «non invocabile la formale applicazione del principio *tempus regit actum*» per escludere la propria competenza a deliberare, ritenendo sussistente un «vincolo di continuazione e di sistematicità» che, congiungendo tutti gli atti compiuti e le opinioni espresse dal senatore Albertini da parlamentare italiano, li ha posti «in diretta connessione teleologica con le prime esternazioni» effettuate quando era parlamentare europeo. Proprio in virtù della peculiarità del caso che stiamo trattando, i senatori democratici esprimeranno dunque il loro voto senza alcun vincolo o indicazione di Gruppo, nell'ambito dei più corretti rapporti fra i poteri dello Stato, esprimendosi liberamente solo e soltanto sulla sussistenza del nesso funzionale, cioè se le opinioni espresse nel caso in questione dal senatore Albertini rientrino o meno nell'esercizio del mandato parlamentare e, pertanto, nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione).*

ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda pensa di far riscrivere le regole della strategia energetica nazionale dagli stessi attori che quegli aumenti stanno determinando. Su questo punto, il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione su cui chiediamo una risposta al più presto. Nello specifico cosa è successo? È successo che il ministro Calenda ha scelto di coinvolgere nella consulenza per lo studio di revisione della strategia energetica nazionale la società privata statunitense Boston Consulting Group, da cui arriva Francesco Cuccia, attualmente capo della segreteria tecnica dello stesso Ministro. Quindi, una persona che ha lavorato alla Boston Consulting Group fino a poco tempo fa adesso è capo della segreteria tecnica, e alla sua *ex* azienda viene conferito questo prestigioso incarico. Insomma, qualche dubbio ci sorge. Sarebbe utile che il Ministro venisse in Parlamento a riferire, invece di affidare a un brevissimo *tweet* le proprie intenzioni.

che questi soldi non li tirerete fuori direttamente attraverso il Ministero dello sviluppo economico, perché non li paga il Ministero, ma li mettono Terna e Snam, quindi, indirettamente, sempre voi italiani. Terna e Snam perché, evidentemente, hanno un futuro legato mani e piedi proprio al destino della strategia energetica nazionale. Quindi, i due attori principali sono quelli che pagano lo studio su cui andrà basata la modifica della strategia energetica nazionale. Tra l'altro, due aziende che prevalentemente sono ad azionariato straniero e, quindi, potrebbero tranquillamente non fare gli interessi nazionali. perché questo studio non è stato affidato i nostri bravissimi tecnici, veramente bravi, presso il Gestore dei servizi energetici, ricerca di sistema energetico e l'ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia, e lo sviluppo economico sostenibile? Perché continuare

ad uno al servizio di interessi particolari privati i cui obiettivi, però, temo non coincidano con un modello di sviluppo sostenibile cui dobbiamo puntare con la strategia energetica nazionale, cioè il raggiungimento dei *target* e degli obiettivi 2030 sulla riduzione delle emissioni,

Penso sia importante ricordarlo anche in quest'Assemblea dopo che in modo ampio e informato è stato ricordato pubblicamente, anche sulla stampa, da Giuliano Amato (che lo volle Ministro nel suo ultimo Governo), Alberto Asor Rosa, Francesco Erbani, Paolo di Paolo, e tanti altri. I motivi per cui penso sia essenziale tener sempre presente il contributo di De Mauro, per me che sono figlia di immigrati del Meridione, venuti a cercare una vita migliore nella grande periferia di Milano, Anzitutto, De Mauro ci ha spiegato che la lingua è un luogo. La lingua, i suoi linguaggi, le sue parole, i suoi lessici sono una grande piazza alla quale si accede e dove si abita. Chi non sa parlare, non sa farsi capire e non capisce, quindi non ha accesso. Non ha accesso ai diritti, non ha accesso alle opportunità, non ha accesso all'emancipazione. Quindi la lingua è un fattore di sviluppo e di uguaglianza. C'è un nesso stretto tra lingua, istruzione e democrazia. In questo primo insegnamento, peraltro, De Mauro ci ha mostrato la sua passione per la conoscenza dei dialetti, per i modi di dire, per i neologismi. Egli svecchiò, anzi forse fondò, la linguistica italiana, ma ne fece una scienza sociale, che esigeva il possesso dei tecnicismi ma poi andava oltre, cercando profondità storica e proiezione futura.

Insomma, per De Mauro la lingua italiana è proprio un "posto bellissimo", in cui possono abitare le città e le campagne, i centri e le periferie, i giovani e i meno giovani. L'altro motivo per cui ricordo De Mauro è collegato al primo e ha un connotato eminentemente politico: la lingua, che è un fattore di sviluppo e di emancipazione, deve quindi contare su una scuola efficace, ricca e stimolante. La sua ultima battaglia, quella sull'analfabetismo di ritorno, nasceva dalla riflessione che la scuola deve insegnare a imparare, a interessarsi sempre di tutto, al gusto della lettura. De Mauro era anche molto ironico, ma la sua ironia era sempre mirata a smontare i luoghi comuni: diceva che leggere è un piacere solo per pochi, più spesso è una fatica, un'operazione intellettuale complessa. Allora ecco che la scuola è un momento fondamentale per l'individuo ma anche per la collettività. La lingua e la cultura sono profili politici. De Mauro spiegava che se, viceversa, dalle conoscenze e dalle capacità acquisite a scuola si regredisce invece di avanzare, ci si perde e si smarrisce la strada per quella piazza così bella che è la nostra lingua, quella stessa lingua in cui è scritta la Costituzione. In un'introduzione a una pubblicazione della nostra Carta costituzionale dell'UTET del 2006, De Mauro esaltava «l'italiano degli italiani», la lingua chiara e profonda in cui sono scolpiti i nostri diritti e i nostri doveri, e dove la dignità della persona è così ben rappresentata.

Signora Presidente, con questo intervento continuo oggi una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Nella notte fra il 26 e il 27 dicembre, a Parma, Gabriella Altamirano, di quarantacinque anni, è stata uccisa a coltellate, assieme a Kelly Manici, transessuale e *drag queen*, dal compagno, che aveva lasciato dopo che lui stesso l'aveva avviata alla prostituzione vivendo dei proventi di quell'attività. Gabriella lo aveva più volte denunciato per atti persecutori e più volte aveva chiamato il 112 perché lui si appostava sotto casa. Salgono così a 33 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno 2016. Molte di loro uccise dopo una separazione, anche solo annunciata. Sempre come reazione ad una recente separazione, si è consumato il 9 gennaio un ulteriore tentativo di femminicidio, a Messina, dove Ylenia Bonavera, di ventidue anni, è stata data alle fiamme dal suo ragazzo ed è ora in ospedale col corpo devastato dalle ustioni. Ylenia non ha denunciato il suo compagno, che anzi ha cercato di scagionare nonostante le prove schiaccianti. Uno schema purtroppo assai consueto, lo stesso per cui proprio ieri una ragazza albanese di si è recata al pronto soccorso di Budrio, nell'area metropolitana bolognese, con un polso rotto dal compagno, che però si è rifiutata di denunciare. Secondo L 'ISTAT, In Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner* o dell'ex *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita, quell'odioso maltrattamento psicologico che consiste nel lasciare che minori assistano ad atti di violenza contro un adulto che, nella gran parte dei casi, è la loro stessa madre. Non si tratta solo di fatti di cronaca. Esistono ragioni culturali profonde della violenza contro le donne e degli atti di femminicidio. Esiste, nel nostro Paese, una questione maschile, intesa come un'incapacità di molti uomini a gestire in modo corretto, paritario e non violento la relazione con l'altro genere. Riproponiamo quindi con convinzione il nostro appello. un appello al Governo, nell'attesa che sia riassegnata la delega alle pari opportunità: la cabina di regia monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, approvata da questo Parlamento in attuazione della Convenzione in Istanbul e, soprattutto, dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. È un appello ai *media*: si smetta di giustificare, anche solo con un linguaggio sbagliato, gli assassini e di colpevolizzare le donne. un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più accettare questa mattanza. *(Applausi)*. Grazie, Presidente.

È stato il primo Ministro della difesa socialista, ai tempi della Guerra fredda ed è stato colui che per primo ha

Accrebbe il bilancio militare, modernizzò l'organizzazione dell'apparato militare italiano, come ampiamente riconosciuto anche in questi anni. Decisivo fu poi il suo contributo anche nelle azioni di soccorso e di ricostruzione, con l'Esercito, in occasione del terremoto dell'Irpinia del 1980.

Ricordo che Mariotti è stato colui che ha creato la sanità che abbiamo adesso in Italia. È stato il padrino della legge n. collocato nel PSI su posizioni autonomiste dove per autonomia, secondo Lagorio, si intendeva autonomia dal Partito Comunista Italiano, il più forte partito della sinistra italiana e il più grande partito partito comunista dell'Occidente. Lagorio sarà sempre a fianco di Bettino Craxi, come lo è stato anche quando questi è dovuto andare in esilio. Concludo

Lui, che era nato in Trentino-Alto Adige, a Firenze ha dato tanto e ha avuto la fortuna di essere tra i collaboratori uno dei padri

Signora Presidente, colleghi, il presente intervento mira a denunziare l'amministrazione scellerata del Comune di Bari da parte del suo sindaco, il caro Decaro, comuni italiani (ANCI). Pensate che per riqualificare il giardino pubblico Isabella d'Aragona nella bellissima città vecchia, il caro Decaro ha fatto abbattere ben 57 pini secolari, tanto da condurre al blocco del cantiere da parte della competente Sovrintendenza. Il fatto, denunciato dalla stampa locale e dal sottoscritto sui *social network*, è stato anche oggetto di un esposto alla procura della Repubblica da parte del capogruppo al Comune del Movimento 5 Stelle, Mangano. Il caso, peraltro, non è il primo ed infatti il caro Decaro, come al tempo da me denunciato, si era già messo in mostra in questa sua veste di *tree killer*, facendo abbattere 18 maestosi pini nel quartiere Japigia, già di per sé depresso, per realizzare delle magnifiche rotatorie in cemento del costo di oltre un milione di euro. A tali imprese va poi aggiunto lo splendido rifacimento della centralissima via Sparano, con la scomparsa di almeno 25 palme, che ormai da anni ornavano la strada pedonale dello *shopping* barese. Potremmo infine ricordare l'assordante silenzio del caro Decaro di fronte alla vera e propria strage di pini compiuta nel luglio scorso all'interno del cantiere per il nuovo parcheggio dell'ospedale pediatrico di Bari.

anche a livello nazionale. Bari è una città con pochissimo verde, eppure il caro Decaro, aspirante tagliaboschi ed ormai affermato *tree killer*, infischiandosene dei diritti alla salute ed alla bellezza dei cittadini baresi e, specialmente, dei bambini, continua inarrestabile la sua vergognosa azione amministrativa, peraltro coadiuvato da un ex parlamentare dei Verdi, già presunto baluardo dell'ambientalismo ipocrita della sinistra, tale Vito Leccese. Insomma un ennesimo squallido esempio di squallore amministrativo di questo PD di Governo. Il Movimento 5 Stelle invita tutti a riflettere sull'importanza del verde nelle nostre città quale inderogabile dovere di ogni amministrazione pubblica verso i cittadini, nel rispetto del loro diritto ad una vita felice e salubre. Per fortuna, signora Presidente, anche per Bari, nonostante il caro Decaro, arriverà presto il momento del cambiamento. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato domani, mercoledì 11 gennaio 2017, alle ore 16,30, per la votazione relativa all'elezione di un giudice della Corte costituzionale. La chiama avrà inizio dai senatori.

Grazie